di Fincantieri di licenziare più di 2.500 lavoratori non possa tenere estraneo il Parlamento, ed il Senato in modo particolare. Mi permetto di richiamare nuovamente l'Assemblea del Senato

Presidente, 2.500 operai sono quasi un terzo della forza lavoro della Fincantieri. Fincantieri ha importantissimo fiore all'occhiello dell'industria italiana. Debbo dire con stupore che in Parlamento non era stata minimamente segnalata una così drammatica accelerazione dell'evoluzione della storia industriale di questo grosso gruppo industriale. Mi chiedo quindi per prima cosa, e dovremmo chiedercelo tutti, con quale lungimiranza queste vicende sono state osservate osservate e sono state considerate. Non credo che davanti ai problemi reali e consistenti della globalizzazione, dello spostamento dei mercati dell'affievolimento di settori industriali la risposta possa essere quella che oggi viene data. C'è un'improvvisa, inaspettata, non annunciata, non contrattata, non discussa con le forze sociali e non discussa in Parlamento indicazione di licenziamento di un terzo della forza lavoro di un grande gruppo industriale. noi siamo in Parlamento e dobbiamo quindi, per prima cosa, indicare una violazione grave di un metodo democratico che deve presiedere sempre a tutte le decisioni industriali quando hanno a che fare con momenti così delicati come quello del lavoro. il nostro Paese possa affrontare la crisi di Fincantieri in assenza di un grande piano industriale del settore e senza

voglio concludere con due osservazioni puntuali su due aspetti che mi sembrano essenziali. Il primo riguarda il ruolo dello Stato: Fincantieri non è un'industria privata ma una società per azioni totalmente posseduta dallo Stato, ed è quindi a quest'ultimo che spetta la responsabilità sia degli indirizzi industriali sia delle indicazioni di gestione al *management* della società. È lo Stato, attraverso il Governo nazionale, che ha la responsabilità di questi elementi. Il secondo aspetto che voglio sottolineare è il ruolo del Governo nazionale in queste circostanze. La questione non ha in questo momento, per quel che riguarda il Partito Democratico, coloriture politiche. Quindi non faccio questioni politiche rispetto al Governo, ma sottolineo che il Capo del Governo e il Ministro dell'economia, che della società ha il controllo in qualità di azionista, debbono occuparsene in modo diretto. In modo particolare, il Presidente del Consiglio deve assumersene personalmente la responsabilità. È incompatibile con lo stato di crisi di Fincantieri che l'attenzione di Berlusconi non sia evidente per il Paese e non sia evidentemente diretta a una vicenda che costituisce ormai una grande questione di Stato. Al *management* di Fincantieri voglio dire che gli amministratori dell'industria di Stato debbono evitare di cadere nel vizio del marchionnismo, cioè di scimmiottare Marchionne. Non c'entrano niente: gli amministratori dell'industria pubblica non sono Marchionne; sono degli organi dello Stato che, per conto dello Stato, debbono amministrare industrie pubbliche. Naturalmente operano nel rispetto del diritto civile, naturalmente debbono tener conto dei vincoli di bilancio, ma anche dell'unico motivo per anche dell'unico motivo per il quale è possibile giustificare la presenza dello Stato in economia, cioè i fini di interesse generale che debbono sempre sovrintendere all'esercizio dell'industria pubblica. La ringrazio, Presidente, e sollecito la Presidenza del Senato a invitare il Governo a venire in

sulla costiera Castellammare di Sorrento è diventata drammatica. Ieri sera in questa Aula ho sottolineato come oggi un congresso internazionale con 3.000 partecipanti non potrà tenersi a Sorrento per il blocco della strada statale sorrentina da parte dei dimostranti. Ciò non significa non essere solidali con i manifestanti che difendono il loro posto di lavoro, ma occorre essere molto chiari su un punto: tutte le manifestazioni sono consentite e libere, ma non quelle che possono provocare un effetto valanga anche in un settore come quello del turismo, in una delle zone più pregiate per il turismo italiano. È vero, infatti, che queste manifestazioni sono da tutelare, ma è anche vero che se si fa ricorso alla violenza

Ieri sera, signora Presidente, ho chiesto alla Vice Presidente di turno di rappresentare al Governo l'esigenza che la riunione convocata dal ministro Romani per il 3 giugno venga anticipata al più presto e si possa tenere a Palazzo Chigi. Pertanto, associandomi a tutte le richieste

sulla crisi della cantieristica, che offriva anche, in modo analitico perché basata su studi e proiezioni e corredata per rilanciare il settore, come hanno fatto altri Paesi dell'Unione europea, venga inserita al più presto all'ordine del giorno. Infatti, la migliore risposta

l'amministratore delegato della Fincantieri è ancora in grado di gestire una crisi di questo genere. *(Applausi

due pattugliatori e, contemporaneamente, il Governo aveva preso l'impegno, attraverso la Comunità europea, di parlare della cantieristica e di riportare in tutto il Paese ‑ quanto sta accadendo a Castellammare si sta verificando in tutte le sedi della Fincantieri

entrati in cassa integrazione fino a quando è stato definitivamente chiuso lo stabilimento. Attualmente, solo 60 operai operano per la manutenzione.

Chiedo al Presidente di far venire subito in Aula il Ministro, perché Castellammare è una città pericolosa. Abbiamo paura che la camorra possa ritornare in quella città,

perché è logico che chi rappresenta enti che ricevono finanziamenti dallo Stato non faccia parte di organismi che dovrebbero indirizzare le politiche dello Stato per questi enti; tuttavia ci sono anche persone estremamente importanti su tutto il territorio, che fanno un lavoro di informazione significativo (che magari ricevono 1.000 o 2.000 euro per un bollettino locale, che ha una funzione importante per le nostre comunità), che verrebbero escluse. Chiedo al Chiedo al relatore che uno di questi due emendamenti sia accolto, e mi auguro che sia il 12.209, che introduce una specie di franchigia: se una associazione riceve un contributo di 2.000 euro, il suo Presidente non può essere escluso dalla competizione per l'elezione ai COMITES. Su questo articolo c'è un emendamento del relatore, il 12.300, al quale presentiamo un subemendamento a firma mia e del senatore Pegorer, il cui testo vorrei consegnare:

alla Presidenza era stato presentato il subemendamento 12.300/2, a firma Micheloni,

Per ricapitolare, senatore Micheloni, di tutto l'articolo 12 e degli emendamenti presentati all'articolo 12 da lei e dai suoi colleghi, restano gli

Con l'emendamento 12.8 si vuole introdurre il meccanismo del voto elettronico tramite posta elettronica certificata. Tale modalità di espressione del voto, già presente in numerosi Paesi europei, è non soltanto più agevole per i cittadini che vogliono esprimere il voto, ma è anche più sicura in termini di garanzia dell'esercizio di voto e di assenza di manipolazioni e dispersioni del voto rispetto a quella per corrispondenza. Mi sembra di avere già assistito più volte a questa manipolazione, ormai appurata; sappiamo che il voto per corrispondenza non arriva mai:

Comitato di chi rivesta cariche presso istituti di assistenza sociale ed enti gestori di attività scolastiche. Le restrizioni del testo proposto dalla Commissione a nostro avviso appaiono esageratamente limitative, restringendo

12.300 credo si illustri da sé, in quanto tende a contenere il numero delle firme per presentare le liste, per permettere una maggior partecipazione di coloro i quali desiderano candidarsi.

perché è breve: "*Dopo il comma 5, inserire il seguente:* «5‑*bis*. Le liste direttamente collegate a gruppi politici che sono presenti in uno o entrambi i rami del Parlamento con almeno tre parlamentari e ne adottano il simbolo ufficiale non abbisognano di suddette sottoscrizioni. Tale limite è ridotto ad uno per le liste collegate a gruppi delle minoranze linguistiche presenti nel Parlamento». è in un punto che avevo cercato di sollevare anche nella discussione generale: ancora pochi minuti fa è stato detto in quest'Aula che questa legge si applicherà in tutto il mondo. Ovviamente non è così, nel senso che la legge italiana si applica sul territorio italiano; questa invece è una proiezione del vigore legislativo italiano in territori dove la sovranità italiana non esiste, quindi c'è un limite massimo alla presunzione che possiamo dare all'attività legislativa da noi realizzata. Avevo detto che la proiezione del vigore legislativo italiano in ambiti territoriali esclusi dalla nostra sovranità - cioè tutti quelli della circoscrizione Estero non sarebbe possibile se nei Paesi terzi non si riconoscesse, più o meno esplicitamente, la coerenza di tali dispositivi che andiamo ad approvare con i principi locali di gestione democratica della *res publica*, cioè della gestione degli

non è consentita: penso in particolare ad alcuni Paesi del Nord-America. Ho già posto il problema in Commissione, e si è trovata una soluzione di compromesso,

non vorrei che l'effetto combinato fosse l'esatto contrario di quanto si paventa dalla stampa specializzata: invece di favorire i gruppi politici nelle elezioni COMITES li si discrimina, in quanto sarebbero gli unici a non poter sottoscrivere le liste, quindi a non potersi presentare nelle elezioni COMITES. Ciò, perché la legislazione locale, che ovviamente è sovrana nei territori

presentato l'emendamento 12.206: non per favorire ma per non discriminare le liste eventualmente collegate a gruppi politici. Ritiro

ho avuto più volte modo di parlare con il collega Micheloni. Io ritengo che dobbiamo escludere dalla possibilità di candidarsi tutte quelle persone che, direttamente o indirettamente, hanno contributi pubblici. Per questi motivi, sono contrario

deliberatamente i partiti dentro questi organismi si rischia di cambiarne la natura, la rappresentanza sociale e l'espressione della ricerca di un consenso. Questa natura è profondamente diversa, perché all'estero le associazioni, anche di opinioni

si tiene una volta per legislatura. È estremamente importante che una volta per legislatura gli eletti di un Paese abbiano l'occasione, prima di tutto di incontrarsi e di avere un quadro

un senso di collegamento e di responsabilità. Il mantenimento di tale assemblea è estremamente importante: spero veramente che il Governo e il relatore accoglieranno questa nostra richiesta. Ritiro

di una organizzazione dello Stato, sia esso centrale che federale, in cui le Regioni, che svolgono una parte importante delle politiche degli italiani all'estero, in posizione paritaria con i Ministeri del Governo centrale, gli assessori regionali ed i rappresentanti degli italiani all'estero, definiscono

di far partecipare una parte di queste organizzazioni alle riunioni del Consiglio generale, ma senza diritto di voto; esse cioè possono intervenire, in sostanza, di istituzioni che stanno a Roma e che devono andare al Ministero degli esteri per partecipare ad una riunione; non stiamo parlando di spostare persone dall'estero o di aumentare dei costi. Si tratta di rappresentanti di enti, organizzazioni e associazioni nazionali che hanno sede

Non me ne vorranno i membri espressione dei COMITES e degli Intercomites, ma a mio avviso possono tranquillamente assicurare la loro presenza nelle sedute di un organo che non è un Ministero. Perciò avrei preferito vederlo soppresso.

è già compreso nell'articolo 5.

vorrei far presente al senatore Micheloni che nulla ha mai impedito, anche durante l'attuale formula del Consiglio generale degli italiani all'esterno, di invitare

che possa essere ragionevole, o procedere con una posizione di maggioranza, naturalmente legittima ma che noi non possiamo condividere. La soluzione di compromesso consiste nel rafforzare la natura istituzionale del CGIE prevedendo una presenza significativa dei presidenti di Regione o degli assessori

mantenendo, tuttavia, il diritto sostanziale di questa rappresentanza ad avere un invito permanente, quindi a far parte del CGIE, sia pure senza diritto di voto. tutto questa componente dal CGIE a noi sembra una soluzione di forzatura, della quale la maggioranza naturalmente si assume la responsabilità, ma che noi non possiamo condividere. Preannuncio che naturalmente il nostro giudizio finale sulla legge dipenderà in parte considerevole anche dall'esito di questo articolo.

28.200, 28.201, 28.202, 28.204 e

32.3 (testo 2)

Presidente, mi spiace che il presidente Tofani, sempre così garbato, abbia usato quest'espressione nei confronti nostri e del senatore Micheloni. Prima di tutto, come il presidente Tofani sa, quando si indicano coperture, molto spesso accade in tanti emendamenti di utilizzare anche questa. detto, il presidente Tofani deve dirci nel merito, al di là della copertura, se è d'accordo sui finanziamenti e sulle proposte che il senatore Micheloni e gli altri firmatari avanzano con questo emendamento, e non pronunciarsi nel merito della copertura che noi abbiamo scelto.

lo spirito con il quale mi sono rivolto al collega Micheloni. Ho parlato di una caduta di tono tile nel senso che abbiamo già discusso di tali questioni, collega. Chiedo scusa qualora si fosse interpretato in maniera ai contenuti, si può anche essere d'accordo, perché il più è sempre meglio del meno; però, dobbiamo fare i conti con la copertura. Questo era l'unico problema.

sono passati, creando (e lo ripeto, come ho già fatto in sede di discussione generale), ancora più confusione. Io mi rammarico che i due punti focali della proposta dell'Italia dei Valori non siano stati capiti e apprezzati, non so se volutamente, anche da parte dell'opposizione. Dato il fine del provvedimento, ossia quello di riformare la disciplina in tema di italiani residenti all'estero, soprattutto nella prospettiva della semplificazione e dell'efficienza degli istituti di rappresentanza degli stessi, scegliere di seguire gli importanti spunti dati dal Gruppo dell'Italia dei Valori avrebbe permesso di addivenire ad un testo - a mio avviso - di gran lunga superiore. La soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero e il trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, non solo avrebbero rappresentato un passo in avanti per il nostro Paese, ma avrebbero anche determinato, e si tratta di un aspetto non trascurabile, un significativo risparmio economico. Ma ho visto che così non si è voluto fare. I COMITES, come anche il CGIE, rappresentano un *unicum*, sono di fatto una anomalia tutta italiana nel sistema istituzionale, comunitario e non. Ad opinione dell'Italia dei Valori, ci troviamo di fronte purtroppo ad un'ennesima occasione mancata. Sono veramente rammaricato, come tutto il mio Gruppo, che non si sia optato per la scelta più utile per il Paese, sia sotto il profilo strettamente funzionale, sia sotto quello squisitamente Ancora una volta, infatti, si sceglie di preferire le lungaggini burocratiche, a discapito del risparmio economico. È ovvio che anche su questo punto l'Italia dei Valori, da sempre contraria ad ogni spreco delle risorse economiche pubbliche, aveva cercato di intervenire. Ovviamente invano! Il testo in esame è la dimostrazione di come questo non sia il modo per migliorare la rappresentanza e l'immagine stessa del nostro Paese e dei nostri concittadini all'estero. Ribadisco che sarebbe necessario ricominciare da capo con maggiore attenzione, con più diligenza, attraverso la predisposizione di un tavolo cui possano sedersi anche i rappresentanti del CGIE e quelli dei COMITES per traguardare una soluzione condivisa, e non una soluzione imposta dall'alto come quella che si realizzerebbe (e

Avendo delle perplessità circa l'affrettata conclusione del provvedimento, vi chiedo di concedermi qualche minuto per esaminare come sia stato affrontato l'argomento in Commissione e come si sia giunti alla sua approvazione. La discussione ha avuto inizio l'8 aprile 2009 con l'illustrazione dei disegni di legge di riforma dei COMITES e del CGIE. Nella seduta successiva successiva del 22 aprile veniva proposta la costituzione di un Comitato ristretto al fine di redigere un testo unificato. Ci sono voluti circa otto mesi perché il suddetto Comitato redigesse questo testo e altri due per iniziare la discussione generale. Poi, l'arresto da parte della Commissione bilancio che, per svariati mesi, non ha espresso il parere sugli emendamenti. Oggi, a distanza di due anni dall'inizio della discussione, ci accingiamo ad approvare modifiche che regolano la vita dei COMITES e del CGIE per renderli, a dire della maggioranza, più consoni ai tempi attuali. Credetemi, non enfatizzo l'approvazione del nuovo testo proposto. Tuttavia, ritengo che questo abbia stravolto completamente la struttura delle leggi riferite ai COMITES e al CGIE. É questo il motivo che mi ha spinto a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma. Analizzando il provvedimento possiamo notare

una netta riduzione del numero dei COMITES che, secondo il mio punto di vista, porterebbe ad una frattura tra rappresentanza di base e territorio, con conseguente possibilità

per renderli quanto più contundenti e incidenti. Infine, si prefigura forse l'abolizione del CGIE. Vorrei spendere qualche parola in più su quest'ultimo punto.

con l'orientamento di gran parte del CGIE e della quasi totalità dei COMITES e accentuerebbe, in modo forse irreversibile, il distacco già evidente verso gli istituti di rappresentanza da parte delle nostre collettività all'estero. Il lavoro in Commissione doveva essere ispirato dalla consapevolezza che gli italiani residenti all'estero sono una risorsa per l'Italia: una risorsa economica, sociale, culturale e politica; ma questo, a mio avviso, non è quello che la maggioranza ha voluto recepire. In Commissione avevamo l'opportunità di dare un segnale forte a tutti quegli italiani nel mondo che ci hanno votato per essere qui. Se ci circondiamo di persone che ci danno fiducia e credono in noi, tutto diventa più semplice: purtroppo, non siamo in grado di trasmettere loro queste garanzie. Come possiamo tranquillizzare i nostri referenti all'estero

tuttavia che «per lo stravolgimento del testo non ci sarà spazio». Questa dichiarazione è stata rilasciata il giorno dopo la conclusione dell'esame in Commissione affari esteri, quando proprio in quella sede si era deciso di rinunciare alla presentazione di proposte emendative e rinviare il testo in Assemblea senza alcuna modifica. Spiegatemi, quindi, il motivo per cui il disegno di legge, calendarizzato in Aula per il 30 marzo, non sia stato approvato rendendosi doveroso il rinvio in Commissione. Ed ancora vorrei capire

«che il provvedimento venga nuovamente affidato all'Assemblea, sussistendo le condizioni per una conclusione dell'esame in prima lettura». Si cambiano posizioni un giorno sì e l'altro anche. Forse l'intento del Governo, con le sue continue e complicate azioni, era quello di affermare la propria volontà scoraggiando così i nostri connazionali. Oggi siamo in procinto di concludere il percorso di questo disegno di legge. Il testo, una volta approvato, passerà alla Camera dei deputati, dove mi auguro che l'argomento venga trattato con maggiore interesse, e soprattutto con una più precisa ed approfondita discussione. Sulla base di quanto

Ovviamente c'è soddisfazione per la riformulazione anche da parte del relatore degli emendamenti degli emendamenti proposti dal nostro Gruppo che riguardano la certezza del voto, evidentemente uno degli annosi problemi che doveva trovare una soluzione. Certamente, non si è arrivati alla perfezione, ma si è sicuramente andati nella giusta direzione, e per questo annuncio il voto favorevole della Lega Nord.

al quale si è anche riusciti a far cambiare idea gli uni agli altri. Il Parlamento dovrebbe essere questo, il luogo dove ci si parla, anche con l'ambizione e la presunzione di convincersi a vicenda e quindi, possibilmente, di trovare insieme le soluzioni migliori. migliori. Naturalmente, quando poi si va al voto finale, bisogna tirare una riga e fare un somma algebrica tra i più e i meno. Ci sono molti più in questa riforma che, vorrei dire, è istituzionale:

degli italiani all'estero, di quella comunità italiana che non è in Italia e che è una delle ricchezze importanti del nostro Paese. Ebbene, questa riforma, che è ancora incompiuta, in attesa dell'esame dell'altro ramo del Parlamento, ha degli aspetti ha degli aspetti positivi, in particolare, quelli relativi alla certezza del voto, e prevede anche un impianto che cerca di essere innovativo rispetto al Consiglio generale, con l'ambizione di dargli nuovo respiro e nuovo ruolo.

alla base degli italiani all'estero; invece abbiamo degli organismi troppo lontani dal nostro punto di vista, perché la soglia per poterli costituire è troppo alta. È previsto un solo COMITES per circoscrizione mentre avremmo preferito un'articolazione più ampia. Poi c'è questa norma sulla

avremmo voluto venisse affrontato in maniera diversa. Mentre abbiamo condiviso la valorizzazione delle Regioni, non possiamo condividere la mortificazione e la sostanziale espulsione dagli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero di tutto quel mondo che fa riferimento all'associazionismo e ai patronati, con norme di incompatibilità sui COMITES e con il rifiuto di prevedere almeno una rappresentanza senza diritto di voto di questi mondi nel Consiglio generale. Per queste ragioni, il nostro voto sarà contrario, sia pure con uno spirito di apprezzamento per il lavoro comune svolto, nella speranza che alla Camera esso possa produrre un risultato perfezionato da portare ai ai nostri italiani all'estero. Essi, infatti, sono una ricchezza fondamentale per il futuro del nostro Paese e possono diventare il nostro *Commonwealth*, la rete

Presidente, sono perfettamente d'accordo sulla prima parte dell'intervento del senatore Tonini, ma ovviamente non sulla seconda.

tutti coloro che hanno contribuito a questo: il relatore, il collega Micheloni e tutti quelli che hanno capito che

avere poi un ascendente sempre maggiore sui nostri connazionali. Credo che il primo tempo sia stato giocato, e su questo noi diamo un

Ricordo che, nella seduta antimeridiana di giovedì 31 marzo, avevano già avuto luogo l'illustrazione e la discussione della mozione e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Mantica, aveva espresso un parere favorevole sull'atto di indirizzo, a condizione che fossero approvate alcune modifiche, che i proponenti non hanno tuttavia recepito nel testo. Nell'auspicio di addivenire ad una soluzione condivisa, i Gruppi avevano successivamente proposto di rinviare il seguito della discussione della mozione. Anche nelle sedute antimeridiane del 13 aprile e del 5 maggio si è convenuto su un ulteriore rinvio. Avverto che il senatore Micheloni ha riformulato la mozione di cui è primo firmatario e che è stato presentato l'ordine del giorno G1 dei senatori Bettamio ed altri.

Lasciare questo tempo necessario vuol dire congelare allo stato le cose, non sulle decisioni future. Se il Governo è rimasto su quella posizione, chiedo di votare il testo 2, con la riduzione della moratoria a 12 mesi.

dall'ordine del giorno che abbiamo presentato. Non si tratta di congelare

Parlamento; a realizzare la prima installazione del Sistema telematico per i Servizi consolari a distanza anche presso il Consolato generale di Londra,

intervenire in dichiarazione di voto? Questo suo intervento assorbe la dichiarazione di voto?

giorno G1, perché se la *ratio* è cercare di razionalizzare i costi, evidentemente, quando ci si trova

pur tenendo conto del motivo principe che ci ha portato a questo lavoro congiunto e a condividere l'operato del collega Micheloni Micheloni e concordando con quanto sottolineato dal senatore Bettamio, la posizione della Lega Nord

palesate dal Governo.

i Paesi nei quali si realizza questa operazione dell'avvenuto cambiamento, abbiamo comprato sedi e stiamo acquistando le attrezzature. Credo che mettere in moto un meccanismo, a metà della cura,

Europa - ma di una razionalizzazione della rete consolare. Sono stati installati 60 sistemi informativi consolari in questo periodo:

Il Governo si apre addirittura su questo, accogliendo un ordine del giorno con cui propone, non di fare un discorso sulle chiusure, ma di approfittare dell'apertura di una nuova sede consolare a Londra per gestire insieme al Parlamento quello che noi riteniamo debba essere il modello del nuovo consolato.

collaborazione fattiva sulla realizzazione di nuovi servizi consolari attraverso l'informatica. Il Governo respinge la cultura della chiusura

in consolati onorari. Alcuni importanti consolati inglesi, compreso quello di Milano, vengono chiusi e si passa a forme diverse di rappresentanza. Aggiungo - devo dirlo con grande chiarezza - che non mi risulta che i cittadini francesi abbiano occupato il consolato francese di Milano mobilitando il consiglio regionale lombardo e parlando male del loro Paese che impedisce loro di avere un consolato. Tutto questo è invece avvenuto nel sistema italiano: abbiamo brillantemente manifestato in tutte le sedi del mondo contro il Governo per la chiusura delle sedi. Credo che anche questo vada riportato all'interno di una norma di rapporti. Non si tratta di chiusure. Giusto per informare, faccio presente che abbiamo chiuso tre consolati in Belgio, che è grande come il Lazio e che aveva cinque consolati.

nonché necessaria, volta, da un lato, a rappresentare e difendere gli interessi del nostro Paese all'estero e, dall'altro, a offrire servizi e tutela alle comunità italiane nel mondo, così da soddisfarne le esigenze. Come noto, i cittadini italiani nel mondo sono circa 4 milioni, ed è necessario che l'Italia si impegni nei loro confronti garantendo l'assistenza attraverso una rete di servizi consolari funzionale ed efficiente. È quindi di primaria importanza che il Ministero degli affari esteri rappresenti e difenda gli interessi del nostro Paese all'estero, offrendo servizi a tutela della comunità italiana nel mondo. Non dimentichiamo che l'organizzazione e la presentazione uffici di rappresentanza all'estero costituisce in molti casi, insieme agli Istituti italiani di cultura, il biglietto da visita del nostro Paese, condizionando sensibilmente la promozione delle politiche del turismo verso l'Italia.

del Gruppo dell'Italia dei Valori peggiorerà sicuramente in modo considerevole la funzionalità di una rete consolare già in forte difficoltà. numerose sono state le critiche e i dubbi espressi in tutte le sedi, comprese quelle parlamentari, da parte degli addetti ai lavori e soprattutto dai rappresentanti degli italiani all'estero. Sono note a tutti le manifestazioni di protesta organizzate dalla comunità italiana in varie città europee interessate dalle chiusure e dalle razionalizzazioni.

La 3a Commissione permanente del Senato ha deliberato all'unanimità la realizzazione di un'indagine conoscitiva che ha come obiettivo quello di conoscere l'effettiva situazione dell'organizzazione dei servizi e della rete diplomatico-consolare italiana del Ministero. Con questa mozione si vuole impegnare il Governo a promuovere nell'immediato uno specifico provvedimento di "moratoria" che differisca per un termine di 12 mesi il piano di ristrutturazione presentato dal Ministero degli affari esteri, a "congelare" la rete consolare nella sua attuale situazione e a tenere conto dell'esito dell'indagine conoscitiva della 3a Commissione. Il fine è quello di addivenire ad un progetto condiviso di profonda riforma della rete e dei servizi consolari italiani nel mondo e di rispettare pienamente i diritti democratici degli italiani residenti all'estero. L'unico punto che l'Italia dei Valori non condivideva, come già ribadito nella seduta del 31 marzo scorso, riguardava la lunga moratoria di 30 mesi, prevista nella prima versione della mozione, perché rischiava di configurare unicamente una scusa per il Governo ad essere inoperativo. Sul punto però abbiamo collaborato e si è addivenuti al termine condiviso di 12 mesi. Per questi motivi, l'Italia dei Valori annuncia il voto favorevole in riferimento alla mozione 1-00379 (testo 2) del senatore

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea del Senato è chiamata ancora una volta ad esprimere il proprio voto su un argomento che, pur essendo sempre di grande attualità, non riesce a trovare una definitiva risoluzione. La mozione del senatore Micheloni invita il Governo a prendere in considerazione l'ipotesi di differire di 12 mesi il piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete consolare. Vorrei ricordare come i consolati, oggi più che mai, svolgano un ruolo fondamentale tra le comunità italiane residenti all'estero, garantendo loro servizi amministrativi, promuovendo lo sviluppo economico, culturale e scientifico. L'Italia ha una vastissima rete diplomatico-consolare che, esclusi gli istituti italiani di cultura, complessivamente annovera 253 sedi (123 ambasciate, 14 rappresentanze permanenti e altre strutture e 116 consolati). Tra i nostri maggiori *partner* comunitari, solo la Francia con 258 sedi (158 ambasciate, 29 rappresentanze permanenti ed altre strutture, 98 consolati) ha una rete complessiva più estesa. Regno Unito, Germania e Spagna, con rispettivamente 233, 221 e 203 sedi, hanno reti diplomatico-consolari di minore estensione della nostra. La rete consolare italiana, con i suoi 116 consolati, primeggia in assoluto ed è quella che determina la nostra complessiva maggiore estensione rispetto a Regno Unito e Germania, che hanno una rete diplomatica ben più estesa della nostra. Ben diverso è il discorso delle risorse umane impiegate: quelle britanniche e francesi, che tra loro grosso modo si equivalgono, sono il doppio delle nostre e quelle tedesche lo sono una volta e mezza. I diplomatici francesi e quelli tedeschi sono circa il 50 per cento in più di quelli italiani e quelli britannici sono addirittura il triplo. Tradotti in termini operativi, dati significano una disparità enorme delle rispettive capacità di occuparsi di settori importanti dell'attività diplomatica.

in capo del personale. Le sue *chances* di svolgere in ciascuno dei settori a lui affidati un lavoro più efficace di quello svolto da due o tre funzionari delle concorrenti ambasciate Francia, Germania o Regno Unito sono poche. Qualche volta ci riesce, ma il più delle volte deve dare priorità ad alcuni settori a scapito di altri. In estrema sintesi, gli apporti aggiuntivi necessari a riequilibrare la situazione sono quantificabili in 1.600 unità, per cento delle presenze attuali, distribuite fra tutte le categorie di personale. Vi è certo una particolare enfasi sul personale a contratto, in linea con le tendenze prevalenti nei Paesi europei presi a paragone: questo, però, è un aspetto che che va attentamente ponderato in chiave di mantenimento di idonei equilibri tra le varie componenti del sistema, secondo i principi condivisi da tutte le organizzazioni sindacali. Anche se accolto nella sua integrità, il prospetto di rafforzamento delle dotazioni del personale non farebbe salire in maniera significativa l'incidenza del nostro bilancio su quello dello Stato. Si passerebbe, infatti, dall'attuale 0,24 per cento allo 0,258 per cento, con un incremento di meno di due decimi di percentuale. A tal proposito, non vedo il motivo per cui si debbano ridurre le sedi diplomatico-consolari. Concludo annunciando il voto favorevole del mio Gruppo e quello dei senatori di

torna all'esame dell'Aula del Senato un tema d'interesse precipuo degli italiani all'estero, solo pochi minuti dopo l'approvazione del disegno di legge di Quella degli italiani all'estero - come già è stato detto - è una popolazione di 4,3 milioni di persone, che ha caratteristiche specifiche, tra le quali mi preme mettere in evidenza il fatto che essa è in continua crescita. Questo fa sì che - lo ribadisco ancora una volta - il totale dei cittadini italiani sia di quasi 65 milioni, non 60 milioni, come viene riportato. Si tratta di un problema particolarmente importante per noi italiani all'estero, molto sentito dalle nostre comunità. comunità. La rete consolare, infatti, ancor più di quella diplomatica, costituisce sempre e comunque un cordone ombelicale con il nostro Paese, il Paese madre. Credetemi, non si tratta di retorica: chiunque parta o emigri lo fa per bisogno, ancora adesso, e così facendo lascia dietro di sé - senza mai sapere bene per quanto tempo - oltre ai propri affetti e retaggi, anche un riferimento statuale che all'estero potrà ritrovare solo nelle nostre propaggini consolari. Ecco perché gli italiani all'estero sono così sensibili al tema della rete consolare. Ed ecco perché, secondo molti di noi, un vero diplomatico (nel senso di un alto ed importante rappresentante dell'Italia al di fuori dei confini nazionali) non è pienamente formato e rappresentativo se non si è degnamente provato in una precedente responsabilità consolare. La ristrutturazione della rete diplomatico consolare all'attenzione di questa Assemblea oggi prevede la chiusura di un certo numero di sedi (particolarmente in Europa) e l'apertura di altre (specialmente in Asia). Qualche settimana fa, di fronte all'originaria versione del testo non avevamo ritenuto di condividerla *in toto* e avevamo argomentato il perché, in quanto rappresentanti parlamentari eletti all'estero, con preferenze espresse ed individuali, da parte degli italiani ivi residenti. Essendo consci e fieri di appartenere ad una Repubblica parlamentare, non potevamo certo accettare l'argomento di trovarci di fronte ad una decisione già presa dal consiglio di amministrazione del MAE, né soprassedere rispetto al fatto che la Commissione affari esteri del Senato ha appena cominciato, seguita a ruota da quella della Camera, una indagine conoscitiva sul funzionamento del Ministero e dunque si vorrebbe avere tempo e modo di approfondire certe situazioni prima di convalidare parlamentarmente certe decisioni. Adesso, mi si consenta di chiarire alcuni punti che differenziano il testo della mozione e dell'ordine del giorno oggi in esame, su proposta dei senatori Bettamio ed altri. luogo, noi italiani all'estero siamo perfettamente consapevoli degli effetti della globalizzazione e di quelli di una crisi, nata finanziaria e sviluppatasi come economica reale, che riguarda tutti i Paesi del mondo. Ne siamo consapevoli perché la viviamo anche di più dei concittadini metropolitani - come li definisce il collega Micheloni, cioè degli italiani residenti in Italia - perché ne subiamo gli effetti in più di un Paese. Siamo anche orgogliosi al riguardo di come il Governo Berlusconi, in particolare attraverso il meritorio operato del ministro Tremonti, ma non solo, abbia gestito la politica economica e di bilancio in tale eccezionale situazione di crisi. Siamo stati critici sull'eccesso di tagli operati rispetto ai capitoli degli italiani all'estero, ma ci rendiamo perfettamente conto, in termini più generali, che la tenuta sociale del Paese sia una priorità rispetto ad altre, pur importanti, considerazioni. Capiamo quindi, per essere chiari, ad esempio, che l'estensione garantita praticamente a tutti della cassa integrazione guadagni nelle sue varie forme possa valere in questi drammatici tempi anche il ridimensionamento di qualche rappresentanza italiana all'estero. Ce ne dispiacciamo, abbiamo fatto del nostro meglio per evitarlo, ma capiamo. Soprattutto, siamo fiduciosi del fatto che con questa barra si riuscirà presto ad uscire dalle secche, tornare a crescere ed espanderci al di fuori dei confini nazionali. Lo crediamo e lo auspichiamo sinceramente, anche perché abbiamo l'ardire di pensare che una maggiore presenza dell'Italia all'estero sia positiva non solo per il nostro Paese e per gli italiani all'estero ma anche per moltissimi altri cittadini del mondo. luogo, il nostro metro di giudizio non è mai stato quello quantitativo bensì quello dell'efficienza. Non crediamo in una onnipresenza dello Stato e rifuggiamo dai suoi retaggi vetero-amministrativi, che si ripercuotono inevitabilmente sulle tasche dei contribuenti italiani. luogo, siamo riformatori, e per questo abbiamo chiesto ed ottenuto la fiducia politica dei nostri connazionali. Siamo quindi d'accordo con lo spirito che anima la ristrutturazione proposta, diretta all'implementazione di una rete consolare più efficiente perché più moderna, in linea con l'evoluzione tecnologica, e meno costosa. A Londra, dove sono emigrato nel 1993 e dove l'influsso della cosiddetta nuova emigrazione professionale ha portato il consolato generale al secondo posto nella classifica delle nostre presenze nel mondo (poco dietro Buenos Aires), con circa 160.000 iscritti, sarà realizzato, in una sede finalmente nuova, un consolato modello proprio in base a questi nuovi e moderni criteri. Ne siamo molto contenti, e vigileremo da vicino sull'implementazione, con l'auspicio di potere presto annoverare molti altri esempi Già la maggior parte dei nostri connazionali ivi residenti interagisce con le locali amministrazioni in via telematica e digitale. Non si vede perché essi non dovrebbero essere in grado di fare altrettanto con una moderna pubblica amministrazione italiana: quella pubblica amministrazione che il ministro Brunetta sta cercando di realizzare con meritoria tenacia. Siamo anche soddisfatti di avere potuto esplicitare le specifiche ed eccezionali esigenze sottostanti l'opportunità di mantenere una presenza consolare a Manchester, nel Regno Unito. In quarto luogo, siamo felici che il Governo abbia recepito nel nuovo testo della mozione la moratoria di 12 mesi: esattamente il periodo che avevamo richiesto (perché giudicato più opportuno rispetto ai 30 mesi richiesti da alcune opposizioni). Dovrà essere questa l'occasione per fare conoscere meglio a noi tutti - ed *in primis* agli italiani all'estero che ne sono tra i maggiori utenti - i criteri e le modalità di funzionamento della grande macchina del nostro prestigioso Ministero degli esteri. *(Commenti del Nessuna ristrutturazione della rete diplomatico-consolare sarebbe, a nostro avviso, degna di questo titolo se si limitasse agli aspetti logistici della apertura e della chiusura di alcune sedi. Anima e cuore della nostra rete sono le persone che a vario titolo ci lavorano dentro, gli interlocutori diretti di noi italiani all'estero, funzionari ed impiegati di ogni livello che, in tutte le parti del mondo, svolgono le loro funzioni col senso del dovere proprio dei rappresentanti istituzionali di un grande Paese: l'Italia. A loro, che sappiamo - a volte - dover convivere con situazioni a vario titolo penalizzanti, deve essere diretta l'attenzione dei ristrutturatori della rete, in modo da garantirne meglio in futuro la dignità, come pure l'efficienza delle loro carriere. In questo ambito, già dalle prossime settimane, proporrò un disegno di legge diretto a promuovere l'utilizzo nelle diverse funzioni amministrativo-consolari (ma anche presso le sedi all'estero delle altre nostre reti nazionali, come l'ICE, gli istituti di cultura, l'ENIT) di personale iscritto all'AIRE, cioè di italiani residenti all'estero. Abbiamo questo patrimonio umano: dopo mezzo secolo - grazie soprattutto all'ex ministro Tremaglia - la Repubblica lo ha finalmente riconosciuto istituzionalmente. Ora cominciamo ad utilizzarlo effettivamente come risorsa del Paese! Per tutti questi motivi, il Gruppo del PdL voterà contro la mozione del pur stimato collega Micheloni e a favore dell'ordine del giorno presentato dall'egregio collega Bettamio e da Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà anzitutto posta ai voti la mozione n. 379 (testo 2) e successivamente l'ordine del giorno G1 per le parti eventualmente non precluse né assorbite.

prevede assistenza e cooperazione attraverso le autorità doganali per garantire l'applicazione delle leggi doganali ed impedire le infrazioni. La finalità è quella di un interscambio commerciale più trasparente e più intenso. L'Accordo include 24 articoli ed è corredato da un allegato. Il disegno di legge di accompagnamento reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, oltre all'entrata in vigore e alla copertura finanziaria, quantificata in circa 30.000 euro. A decorrere soprattutto dal 2011, tale onere legato ai previsti scambi di funzionari, ai costi delle indagini su specifiche infrazioni doganali, alle disposizioni di testimoni ed esperti e alle eventuali riunioni della commissione mista.

parere conforme a quello del relatore.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta,

nella *Gazzetta Ufficiale.* DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo

questo Scambio di lettere dispone la cessione alla FAO di alcuni locali di Palazzo Blumenstihl, che è del demanio, destinati ad ospitare il segretariato della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, attraverso l'aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990. Ci sono alcuni oneri di manutenzione derivanti da questo Scambio di lettere: in particolare, l'onere viene quantificato in 200.000 euro annui a decorrere da quest'anno. Tali oneri comprendono la quota di spese di manutenzione di questi locali di Palazzo Blumenstihl e il contributo italiano al bilancio della Commissione stessa, che è di pari importo e corrisponde al 6,17 per cento di detto bilancio. Altri Paesi si erano offerti di ospitare questa Commissione, tra cui Malta e la Spagna, ma i Paesi membri della Commissione (che sono gli stessi membri della FAO) hanno preferito Roma per le possibili sinergie ed economie di scala derivanti dalla prossimità alla sede della FAO. Pertanto, signor Presidente, proponiamo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Chiedo

lo ha fatto sia al Vertice FAO che al G8). Rispetto a quei milioni di euro, in fondo, questo costituisce un impegno minimo. Anzi, speriamo

con i pagamenti che riguardano la lotta alla fame del mondo e la difesa dell'alimentazione. In ultimo, segnalo che proprio su questi temi è stata presentata dal Partito Democratico, in particolar modo dalle colleghe Bertuzzi e Pignedoli, una mozione che riguarda le questioni di pane e democrazia aperte nel Maghreb e nel Nordafrica, che non sono nate per caso ma da precise situazioni agroalimentari che riguardano demografia e alimentazione. Su questi temi, oltre che sull'affitto dell'immobile, cui siamo favorevoli, e sull'impegno nei confronti della FAO, vorremmo che il Governo italiano fosse disponibile.

Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo può essere sicuramente considerato un successo dell'Italia, raggiunto qualche anno fa per la verità, al termine del precedente Governo Berlusconi, quando l'Italia riuscì a battere altre due importanti candidature, come ricordava il presidente Dini poc'anzi, rappresentate da Malta (che all'epoca aveva il Commissario europeo per la pesca,

per tale organismo, come siamo lieti che il Ministro delle politiche agricole abbia indicato, con il pieno consenso di tutte le organizzazioni della pesca italiana, il professor Cataudella, un insigne biologo marino italiano, quale presidente di questa importante istituzione che da oggi potrà essere operativa nella nostra capitale. Quindi, visto che all'epoca partecipai partecipai a quel lavoro con la massima determinazione, saluto questo rinnovato e importante successo del nostro Paese. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che eventuali ulteriori spese relative all'ubicazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) non siano a carico del bilancio dello Stato».

voto favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord. nella *Gazzetta Ufficiale*. DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959,

provenienza necessitava di una apposita richiesta dello Stato medesimo di trasferimento del detenuto. Solo in questi casi si può procedere anche senza il consenso del condannato. Anche in seguito all'incontro svolto il 10 gennaio 2011 tra una rappresentanza della nostra Commissione

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, osservando tuttavia la necessità di tenere in considerazione la disciplina, approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 4262) concernente l'istituzione di squadre investigative sovranazionali, al fine di evitare una legislazione contraddittoria in relazione agli oneri con gli accordi che il Paese stipula in relazione a questo tema». Senatore Pedica, a ratificare questo Accordo. Sostenere la collaborazione giudiziaria, la trasparenza delle relazioni tra i Paesi e l'efficacia della tutela dal crimine delle nostre comunità è infatti fondamentale soprattutto a tutela della sicurezza collettiva. ben garantirà una maggiore efficacia nell'attività investigativa tra le polizie e le magistrature dei due Paesi, nonché favorirà l'estradizione ai fini dell'espiazione della pena sia dei cittadini italiani nel Paese albanese che viceversa. Per questi motivi annuncio

i tantissimi docenti precari che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio hanno ottenuto delle ordinanze sospensive di un provvedimento che li avrebbe visti inseriti in coda alle graduatorie, non sulla

insegnanti. È successo che sono stati nominati commissari *ad acta* per dare esecuzione a queste ordinanze sospensive del TAR Lazio che stanno comunque esercitando il loro ruolo facendo gli inserimenti e modificando le graduatorie provinciali. Tuttavia, lo stanno facendo illegittimamente, perché quel provvedimento del TAR

soprattutto in paradisi fiscali come le Cayman, e che per ripianare le perdite molti di essi dovranno dismettere il patrimonio immobiliare, creando grandi problemi agli inquilini e a coloro che non si possono permettere di acquistare un immobile. Per quanto riguarda l'ENPAM,

rispondesse puntualmente alle interrogazioni forse riuscirebbe a prevenire fenomeni di *mala gestio* che possono mettere a rischio il risparmio previdenziale di migliaia di iscritti, come nel caso di specie. Mi perdonerà, signor Presidente, se continuerò a porre questi problemi ma il sudato risparmio previdenziale non può essere messo a repentaglio da investimenti a rischio in titoli tossici, soprattutto nelle isole Cayman. *(Applausi

Senatore Pedica, non so se quanto dice lei corrisponda esattamente al vero. Se dovesse essere così, le assicuro che ciò costituisce un fatto molto grave, e lei sa benissimo che il Parlamento, tutelando lei in questa posizione, tutela anche la sua funzione.

sull'avvocatura dello Stato affinché solleciti il TAR a ritirare la nomina dei commissari. Infatti, dopo che il TAR ha dichiarato la propria incompetenza